che, per l'importo che abbiamo citato (3,4 miliardi), andrebbero a bloccare completamente il sistema dei tribunali. Diamo anche un suggerimento: se decidete di non accogliere il nostro emendamento, fatevi almeno promotori

a danno delle imprese aggiudicatarie di appalti di dispositivi medici, mentre nella peggiore delle ipotesi - mi permetta il Governo - rappresenta una tangente legalizzata. Il Governo ha deciso di far finanziare alle imprese aggiudicatarie di appalti di dispositivi medici il cosiddetto governo dei dispositivi medici, un meccanismo di cui ancora sappiamo molto poco. si tratta di un costo in più per le imprese aggiudicatarie di appalti nel settore della sanità che andrebbe inevitabilmente a ricadere sul costo finale dei dispositivi in questione e perciò sul Sistema sanitario nazionale, che pagherebbe in ultima analisi le spese di una misura miope. In più, questa modalità di finanziamento della *governance* dei dispositivi medici da parte dei privati è in totale antitesi con la *mission* di questo organismo, perché andrebbe ad alimentare andrebbe ad alimentare un rapporto poco trasparente e torbido tra controllore e controllati, in quanto i grandi *player* del dispositivo medico diventerebbero i principali finanziatori del sistema che dovrebbe controllare la trasparenza delle gare d'appalto a cui partecipano. Con l'emendamento 15.15 chiedo quindi al Governo di abrogare questo meccanismo che evidentemente condurrà a un conflitto di interessi palese e non potrà quindi sortire effetti virtuosi. Fermatevi - lo dico al vice ministro Sileri - questa cosa è gravissima, non potete far finta di niente.

Grazie

direttiva sull'insolvenza delle imprese. La direttiva impone agli ordinamenti nazionali una semplificazione degli istituti per l'insolvenza, che porterebbe a grandi benefici sia per gli imprenditori che per l'efficienza della giustizia. In Italia abbiamo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che regolamenta la materia, ma che, a nostro avviso, soprattutto in questo momento storico va cambiato e riadattato a ciò che ci chiede l'Europa. L'approccio della direttiva, infatti, è molto liberale, mentre la regolamentazione prevista dal nostro codice presenta aspetti di marcata statualità. La loro applicazione, inoltre, rischia di condurre a liquidazione certa un numero elevatissimo di imprese che si trovano in situazione di crisi a causa dell'emergenza sanitaria. Faccio l'esempio della procedura dell'allerta attivabile per sostenere l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi. Nella direttiva la procedura può essere attivata solo dall'imprenditore, mentre nel codice italiano la procedura di allerta può essere attivata non solo dall'imprenditore, ma anche da soggetti come l'INPS o l'Agenzia delle entrate. È chiaro, quindi, che l'attivazione della procedura da parte di quest'ultimi determina perciò solo un effetto dannoso per l'imprenditore che si troverà a essere automaticamente monitorato e messo sotto la lente di ingrandimento. Di conseguenza, non è difficile immaginare che avrà ancora più difficoltà a rimanere a galla. Con l'emendamento 20.0.38 chiedo due cose: innanzitutto la modifica della disciplina italiana, molto più rigida di quella europea, per adeguarla e allinearla alla direttiva sull'argomento, che è molto più liberale; luogo, chiedo di posticipare la data di entrata in vigore della procedura di allerta di un anno fino al 1° settembre 2022, per evitare che troppe imprese possano essere esposte alle procedure di crisi praticamente in automatico, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo in cui effettivamente molte aziende si trovano in difficoltà economica.

Signor Presidente, i primi sei mesi dell'anno con la presenza della grave pandemia e della crisi che ne è derivata hanno messo in secondo piano un fatto rilevante: lo Stato continua a non pagare i propri fornitori. Lo dico al Governo con cui abbiamo cercato in tutti i modi di interloquire e di farci comprendere. Non ve lo stiamo chiedendo noi, ma i cittadini: pagate le imprese e i debiti dello Stato alle imprese, tanto più in una circostanza come quella che stiamo vivendo dove dite che mettete a disposizione ristori immediatamente. (*Applausi*). Non si capisce quale contraddizione riuscite a giustificare non affrontando questo problema. aggiungo che il 28 gennaio di quest'anno la Corte di giustizia europea, con la sentenza che ho tra le mie mani, ha condannato la Repubblica italiana e lo Stato. Leggo direttamente dal dispositivo la Corte di giustizia dichiara e statuisce: «Non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni»

abbiamo presentato emendamenti che prevedono in maniera molto semplice e precisa di assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti dagli articoli 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativi alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; rafforzare e dettare precise indicazioni al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione; determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento dei costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva. Quello che abbiamo scritto qui dentro è pedissequamente quanto prevede la sentenza della Corte di giustizia europea. Rappresentanti del Governo, questa non è un'opinione politica, è un dovere, un obbligo che ha lo Stato nei confronti dei fornitori e a tutt'oggi siete insolventi e soprattutto nascondete ai cittadini la verità. Porto tutto questo all'attenzione del Ministro: se oggi entrate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze vi apparirà una schermata aggiornata al 5 ottobre 2018, da cui risulterebbe

Richiamo il Governo alla necessità di approvare questo emendamento e di pagare definitivamente i debiti che lo Stato ha con i propri fornitori.

ove non possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva UE 2019/904, prevedere la graduale riduzione del consumo dei medesimi entro il 2026, consentendo l'immissione sul mercato di tali prodotti qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile»; 2) *alla lettera c) sostituire le parole* «dall'uso» *con le seguenti* «dal rilascio».

con prodotti chimici. Invito dunque il relatore a un ulteriore approfondimento, perché stiamo proponendo qualcosa in contrasto con la direttiva stessa.

Chiedo al relatore se deve ulteriormente riflettere su quel problema relativo all'articolo 15.

La seduta è ripresa. Chiedo al presidente Pesco di aggiornarci rispetto al lavoro che sta svolgendo la 5a Commissione permanente e chiedo altresì, visto che siete ancora in seduta,

Informo che la 5a Commissione ha espresso il parere sugli emendamenti 15.100 (testo 2) e 22.103 (testo 3).

*segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 15.100 (testo 2), Costituzione. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemb1ea, sulla proposta 22.102 (testo 3) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: con il seguente: destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione sul mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo

Presidente, ho riformulato il mio emendamento per cercare di andare incontro alle istanze e alle richieste del Governo e della maggioranza.

fossi convinta della giustezza della riformulazione stessa, per cercare di andare incontro alle esigenze e alle istanze della maggioranza e del Governo, nonostante - lo ribadisco

andrà a supervisionare i controllati da cui sarà finanziato: in sostanza, l'organismo controllerà i controllati che lo finanzieranno cioè, le aziende aggiudicatarie degli appalti. A me sembra una cosa folle e vergognosa. Mi auguro, pertanto, che il Governo almeno nella prossima legge di bilancio ponga un rimedio e sani questo *vulnus* tremendo che si sta creando e che ovviamente sarà fonte di meccanismi torbidi e poco trasparenti tra quell'organismo e le imprese, le grandi *lobby* dei dispositivi medici, perché questo è innegabile. Mi appello quindi al Governo

Signor Presidente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 2017, ha stabilito che la maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 12193 del 2019, ha confermato le statuizioni della Corte costituzionale. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 - come ben sappiamo - vieta e punisce come delitto l'utero in affitto. Questa stessa Aula del Senato, in data 22 novembre 2018, ha approvato una mozione nella quale si leggeva che l'utero in affitto è da considerarsi a tutti gli effetti come violenza contro le donne. Non capisco, quindi, per quale ragione sia stato formulato un parere negativo

il rispetto dei diritti inviolabili della persona e il diritto alla dignità umana. Chiedo, quindi, che il Governo e il relatore rivedano il loro parere negativo e che questa Aula si si pronunci a favore dell'ordine del giorno, che non farebbe altro che ribadire, anche nel contesto europeo, ciò che il nostro Paese sostiene e che è perfettamente in linea con la

mi preme sottolineare la nostra posizione nettamente favorevole all'ordine del giorno G15.100. Anche noi ci auguriamo, come il collega Pillon, che il Governo possa rivedere questa posizione. Quest'ordine del giorno è in linea con quanto quest'Aula ha già approvato - come menzionato dal senatore Pillon nel suo intervento - ed è sicuramente in linea con una proposta di legge di Fratelli d'Italia, che

posizione, perché riteniamo che questa pratica sia svilente della dignità e dei diritti umani; che si consumi sul corpo delle donne; che sfrutti le condizioni di povertà e che, in una parola, si traduca in acquisto e, quindi, mercificazione dei bambini. In questa nostra visione della vita e del mondo, il nostro voto favorevole all'ordine del giorno in esame sarà netto e convinto.

che ovviamente sfrutta la donna ma che è già vietata in tutta Europa, è forse più funzionale a un gesto di

mi ero ripromesso di parlare nel caso che il Governo o il relatore non avessero dato spiegazioni al loro parere contrario. Posso parlare sulla fiducia: non ci sarà spiegazione, perché c'è la pessima abitudine di non dare spiegazione su niente,

condanna di una pratica che riduce la donna a strumento di produzione di beni da vendere, e i beni da vendere sono dei bambini, degli esseri umani. Se non c'è contrarietà su questo, allora il parere sia favorevole. Oppure si ha paura di disturbare qualcuno? Si ha paura di ostacolare un disegno di legge che sta andando avanti alla Camera? alla Camera? Ce lo spieghino. Noi voteremo a favore, perché per noi i bambini non sono merce e le donne non sono uno strumento di produzione.

dopo questo invito caloroso, vorrei apporre la mia firma Presidente, per il rispetto che porto nei confronti di tutte le colleghe

nel rapporto tra il Parlamento di una Nazione e le istituzioni europee. Dovremmo evitare, per quanto possibile - e abbiamo cercato di farlo - di immettere in questo veicolo legislativo di recepimento di 33 direttive europee questioni che, per quanto legittime

quest'ordine del giorno sarebbe stato dichiarato inammissibile. *(Applausi)*. Visto che è stato ammesso, il nesso c'è. Caro relatore, è attinente alla materia, quindi va votato; assumetevi la vostra responsabilità e votate "sì" o "no" nel merito.

In premessa, devo salutare la nomina del collega Licheri a Presidente del Gruppo. Me ne rallegro, ne sono felice. Di solito un applauso si fa, ragazzi! Sono convinto che con lui come Capogruppo ci divertiremo molto e ci sarà un'aria frizzante. Il richiamo al Regolamento è il seguente: il collega Licheri o si astiene o vota a favore dell'ordine del giorno; oppure, essendo intervenuto in senso contrario il collega Airola,

ritengo che questa tematica così difficile non possa essere trattata qua, nell'ambito di un ordine del giorno, presentato su un disegno di legge che non c'entra tanto. Semmai, ci dev'essere una discussione approfondita. Ai colleghi di destra, che adesso si preoccupano tanto per il corpo delle donne, vorrei ricordare che sono loro, a distanza di

Grazie

molto all'attualità e chiede al Governo di impegnarsi a tenere conto della Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 nel pieno rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, con riferimento alla sicurezza dei vaccini e ai possibili effetti derivanti dalla loro somministrazione. È importante che si aderisca alla Strategia europea per i vaccini contro la Covid-19 ed è fondamentale che ci sia una piena adesione del nostro Paese e che parallelamente siano rispettati i diritti costituzionali.

Ritenevamo essenziale inserire in questa legge di delegazione, per coerenza, per opportunità, ma soprattutto per rispetto dei lavoratori e delle imprese italiane, l'abrogazione immediata della cosiddetta *plastic tax*, all'articolo 1, comma 634, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019, o quantomeno la sua eliminazione per le categorie di prodotti alimentari comunemente percepite come essenziali. Come questa recente emergenza sanitaria ci ha dimostrato, la possibilità di garantire al consumatore approvvigionamenti costanti e durevoli nel tempo è strettamente legata al ruolo degli imballaggi plastici moderni, che con un ridotto contenuto di plastica consentono di applicare le opportune tecnologie industriali, le quali, senza alterare le caratteristiche nutrizionali e organolettiche degli alimenti, ne garantiscono durabilità e sicurezza igienico-sanitaria,

capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti, dobbiamo ancora assicurare gli imballaggi in plastica. Non ci siamo svegliati

insieme fatturano 35 miliardi di euro e danno lavoro, tra dipendenti diretti e indotto, a 100.000 persone. A questo aggiungiamo anche tutta la filiera di Federalimentare.

i milioni di banchi acquistati con i bandi approvati dal Ministero dell'istruzione, a firma del commissario Arcuri, e utilizzati nelle scuole sono interamente di plastica? *(Applausi)*. non prendiamoci in giro. Aboliamo definitivamente la *plastic tax* e permettiamo ai nostri produttori di produrre, come stanno facendo, ma senza costi aggiuntivi. Votiamo convintamente a favore di questi emendamenti, a nome di migliaia di imprese e di lavoratori italiani,

la verifica del numero legale)*.

sull'emendamento precedente ci siamo astenuti, perché abbiamo preso atto di uno sforzo da parte del Governo. Diamo atto

Consentite però di introdurre quei prodotti, solo se in plastica biodegradabile e compostabile. È giustissimo: anche noi siamo a favore e a sostegno di un comparto,

bioplastica, se trattata chimicamente, al pari della plastica: questo non l'avete ricordato. Nella foga ideologica di adottare questa direttiva, c'è stato un errore, con l'emendamento approvato, a prima firma della collega Floridia. Dunque l'emendamento 22.104, ora in esame, vuole

ci asterremo. Si maschera dunque, con una definizione che illustra un errore di traduzione nel testo italiano, che parla di "tazze" e non considera i bicchieri, quello che in realtà era stato un intervento punitivo apportato da un altro emendamento, approvato dalla maggioranza. In conclusione,

a 22.0.211. Colleghi, per dare continuità nello svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e in considerazione del fatto che l'informativa del ministro Lamorgese è prevista a partire dalle ore 17, la Presidenza

L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sui recenti disordini accaduti in alcune città italiane».

Signor Presidente, onorevoli senatori, la complessiva situazione socio-economica del Paese risente della diffusione dell'epidemia, che sta assumendo una valenza totalizzante nello scenario nazionale e internazionale, con riflessi inevitabili anche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, specie in questa fase, in cui è ripresa la crescita dei contagi. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che le misure emergenziali, sia quelle governative sia quelle disposte dalle Regioni in relazione alle specifiche esigenze dei territori, hanno determinato per la generalità degli italiani, soprattutto per alcune categorie particolarmente colpite. Ho già detto - e lo ribadisco anche oggi, qui - che il Governo è in costante ascolto delle voci di disagio e per tale ragione, già a partire dalla scorsa primavera, sono stati messi in campo interventi a supporto dei lavoratori e delle categorie maggiormente in sofferenza, con l'obiettivo di intercettare per tempo i fattori potenzialmente idonei a generare criticità nelle famiglie e nei contesti produttivi e ciò anche con lo scopo di prevenire possibili infiltrazioni criminali nell'economia legale e il conseguente aumento del rischio di usura. In questa direzione, già ad aprile, ho dato avvio a un'attenta attività di monitoraggio degli esiti socio-economici della pandemia, attivando i prefetti, e di recente ho richiesto un quadro aggiornato della situazione. A seguito dell'inasprimento della curva pandemica e delle nuove misure di restrizione adottate, è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri il cosiddetto decreto ristori, che, con uno stanziamento di 11 miliardi di euro, ha disposto interventi a sostegno dei settori più coinvolti dall'applicazione delle restrizioni imposte con l'ultimo In tale difficile contesto, accanto alle civili proteste di cittadini e lavoratori per le nuove e più restrittive misure, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza e di guerriglia urbana, connotati da atti di vandalismo e da veri e propri saccheggi. Si è trattato di episodi che hanno trovato nelle ragioni del malcontento soltanto un occasionale pretesto. Lo conferma il fatto che tutti i vari episodi di violenza accaduti nelle varie piazze d'Italia hanno visto all'opera soggetti che nulla hanno a che fare con le categorie interessate dall'applicazione dei provvedimenti governativi anti Covid. È stato infatti accertato che a tali manifestazioni hanno partecipato, in maniera preponderante, frange violente riconducibili a vari e distinti ambiti, che vanno dai movimenti di estrema destra ai centri sociali, uniti dalla tematica negazionista, fino a ricomprendere i settori più estremi delle tifoserie. Non è da sottacere il contributo di frange giovanili, conseguente al rinnovato attivismo negli ambienti studenteschi, e di una componente violenta di disagiati sociali, composta anche da extracomunitari che si inseriscono nella protesta per mero tornaconto personale, come avvenuto negli scontri di Torino e di Milano del 26 ottobre scorso. Il momento di contatto tra questa componente oltranzista e i legittimi manifestanti è avvenuto nella maggior parte dei casi attraverso i canali *social*, che hanno garantito l'immediatezza e la diffusività delle informazioni relative alle previste iniziative. Le caratteristiche del *social* favoriscono infatti inevitabilmente l'estemporaneità delle manifestazioni pubblicizzate da parte di singoli individui o gruppi non sempre strutturati e non rispondenti ad una strategia unitaria ma accomunati soltanto da finalità antigovernative. Nello svolgimento degli eventi anche l'elemento della territorialità ha un ruolo rilevante per la specificità di alcuni contesti sociali. Nel caso di Napoli, realtà da dove sono partite le proteste lo scorso 23 ottobre, le forti limitazioni imposte hanno avuto un impatto anche sul terreno della piccola criminalità. Diverse sono le segnalazioni pervenute in questi giorni dalla rete delle prefetture sulle manifestazioni da parte di categorie maggiormente colpite, che a partire da Napoli hanno determinato momenti di tensione anche in grandi realtà come Torino, Roma e Milano. A Torino, nella serata del 26 ottobre scorso, hanno avuto luogo nel centro della città due manifestazioni, una in Piazza Vittorio (con circa 1.500 persone) l'altra in Piazza Castello (con circa 1.000 persone), con la presenza di frange *ultras* della Juventus e del Torino. Sia in Piazza Castello sia nei pressi della sede della Regione si sono verificati lanci di bottiglie, pietre e bombe carta all'indirizzo delle Forze dell'ordine. A tali episodi hanno fatto seguito danneggiamenti e saccheggi presso numerosi negozi del centro cittadino (40 gli esercizi commerciali coinvolti) e atti vandalici nei confronti di auto parcheggiate e mezzi delle Forze dell'ordine. A seguito di tali fatti, dieci persone sono state tratte in arresto, due sono state denunciate, mentre risultano feriti dieci operatori delle Forze di polizia. A Milano, la sera del 26 ottobre, un gruppo di circa 400 persone, tra cui appartenenti all'area anarco-antagonista milanese un folto gruppo di giovani, nonché soggetti del mondo del lavoro autonomo, ha provocato vari danni, costringendo le Forze di polizia a condurre brevi cariche di alleggerimento e lancio di lacrimogeni. Da una prima analisi dei fatti, emergono delle peculiarità nelle proteste del capoluogo lombardo, quale l'età dei manifestanti: delle 28 persone denunciate per danneggiamento e violenza, 13 sono minorenni. A Roma, dopo le manifestazioni del 24 ottobre, si sono registrate nella serata di ieri tre diverse iniziative di protesta rispettivamente in Piazza Cavour, in Via XX Settembre (regolarmente preavvisata dalla categoria dei tassisti) e in Piazza del Popolo (pubblicizzata su Facebook da compagini di estrema destra). Ovviamente, per tutte le manifestazioni sono in corso le attività investigative con il coordinamento delle competenti autorità giudiziarie, al fine di individuare i responsabili delle violenze. Stamattina si è svolto il Comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica e vi è stata in quella sede un'approfondita analisi dei fatti all'esito della quale hanno trovato piena conferma le immediate risultanze investigative. Desidero quindi assicurare al Parlamento che la situazione del Paese è seguita con la massima attenzione e che terremo in considerazione ogni minimo segnale di allarme perché la protesta non venga a turbare ulteriormente un clima già profondamente scosso dalle conseguenze della seconda ondata pandemica. Il bene comune è tenere insieme il Paese in questo momento e respingere ogni tentativo di aizzare la protesta e di alimentare derive ribellistiche. L'obiettivo comune deve comunque essere quello di assicurare la tenuta sociale del Paese, da un lato con l'impegno profuso dal Governo anche in queste ore di garantire risorse adeguate alle famiglie e alle imprese più esposte nell'attuale contingenza economica e, dall'altro, attraverso una ferma ed efficace azione di contrasto delle azioni violente tesa a garantire la sicurezza di tutti nel pieno rispetto della libertà costituzionale e di manifestazione del pensiero.

sono singoli episodi che vengono portati all'attenzione a livello territoriale. Ciò emerge dalle indagini fatte e dalle evidenze che risultano agli organi di Polizia.

la sua relazione corrisponde a un dovere istituzionale per il quale la ringraziamo perché con la sua informativa oggi ha dato esatto a quest'Assemblea di come i professionisti del disordine pubblico e della cieca violenza hanno oscurato il tentativo legittimo di migliaia di commercianti, di lavoratori e famiglie di manifestare un dissenso rispetto a scelte, condivisibili o meno, che le istituzioni devono inevitabilmente prendere per evitare l'aumento dei contagi e dei ricoveri. I teppisti che in questi giorni hanno messo a ferro e fuoco Napoli e tante altre città italiane aggredendo Forze dell'ordine e giornalisti devono essere perseguiti e assicurati al più presto alla legge. La stragrande maggioranza dei napoletani è composta da persone oneste di grande dignità, lavoratori, gente altruista e generosa, persone dedite alla famiglia e al prossimo e rispettose delle leggi, che non meritano di essere criminalizzati per colpa di una banda di delinquenti.

Fatta questa doverosa premessa, dopo i fatti di questi giorni, mi chiedo perché allora in questo momento non stiamo tutti insieme a fronteggiare la crisi che sta diventando un fuoco nelle città. Credo sia necessario, mai come oggi, attivare un clima di concordia nazionale perché il vicolo cieco in cui ci ha gettati la pandemia impone la piena condivisione delle responsabilità e l'ascolto a ogni livello istituzionale. Questo fuoco che brucia nelle piazze si può domare soltanto con risposte adeguate e interventi concreti che non rincorrano continuamente gli eventi ma che li prevedano con largo anticipo. Ci aspettano ancora settimane intense e difficili. Bisogna convivere con il coronavirus; dobbiamo arrivare al vaccino vaccino e distribuirlo bene. Dobbiamo organizzare una logistica per il vaccino che sia esattamente l'opposto della gestione logistica del tampone. Se stiamo vivendo una stagione d'emergenza allora è sacrosanto e doveroso che l'Italia acceda ai 37 miliardi di euro del MES per consentire quella sicurezza sanitaria che è alla base della nostra sicurezza economica. Potremo agire sulla sanità, sui trasporti, sulla medicina territoriale e su tutte quelle criticità che non hanno consentito di tenere sotto controllo questa seconda ondata. Lo dobbiamo fare nel nome di questo nuovo stop che il Presidente del Consiglio ha chiesto agli italiani e che davvero potrà portare a conseguenze nefaste ed irreversibili. Caro Ministro, condivido il suo appello ai cittadini onesti di isolare i violenti, ma facciamo in modo che la convivenza con il virus non diventi un incubo per tutti i lavoratori della cultura e dello sport, della ristorazione, del settore dei congressi e degli eventi, delle agenzie di viaggio, degli stagionali, dei liberi professionisti, degli artigiani che avevano fatto tutti gli investimenti necessari per riaprire in sicurezza. Non dobbiamo pretendere di essere autosufficienti. Abbiamo il diritto, anche se all'interno della maggioranza, di pretendere decisioni concrete, rapide e più condivise. Lo pretendiamo nei confronti di un Paese che si è sacrificato e che, di colpo, è colto dal dubbio di averlo fatto inutilmente. Noi di Italia Viva siamo al Governo non per cullarci in un esercizio di autocompiacimento ma per evitare che errori e ritardi gettino il Paese in una spirale di violenze e disordini da cui sarebbe difficile tornare indietro. nei primi sette mesi del 2020 assunzioni in calo del 42 per cento. Unioncamere: 44.000 nuove imprese in meno durante il *lockdown*.

si insinua tra le piccole e medie imprese, nel 2019 segnalate 105.000 operazioni di riciclaggio e i dati sono sempre in aumento. Nel settore terziario 40.000 imprese rischiano l'usura. Dove non arrivano le banche arrivano le mafie Era chiaro a tutti che la situazione esplodesse, signor Ministro, e che i cittadini non potessero reggere una situazione dove il conto delle ingiustizie fosse per lo più a loro carico. Per quanto ancora sopporterete il pianto di cittadini per bene, piccoli imprenditori che costringete alla chiusura, lavoratori senza cassa integrazione e con la paura di essere licenziati? Famiglie al verde, anche per bollette salatissime che non sapete tagliare. Per quanto tempo sopporterete questa disperazione? Un virus globale sta facendo saltare anche la globalizzazione con tutto il suo carico di ingiustizie e le ingiustizie, dopo un po', si riversano nelle piazze. I lavoratori della Whirlpool si riversano in autostrada perché nessuno ha voluto difendere le loro ragioni, sacrificate allo strapotere violento di una multinazionale che può calpestare i diritti del lavoro ed andarsene. Lo stesso accade dove il padrone multinazionale umilia la vita dei cittadini. Avete pensato alle piazze in termini virtuali o in termini liquidi? Le periferie senza servizi, tagliati in nome delle politiche di austerità, diventano infatti periferie liquide, invisibili. Il controllo del territorio è stato dimenticato o sacrificato perché tanto poi ci pensano le belle parole o le frasi di circostanza, che anestetizzano la questione. «La violenza va condannata» è una frase giusta in sé, ma che perde fibra se chi devi rimuovere le cause che l'alimentano non fa nulla per rimuoverle. Davide si ribellerà sempre contro Golia con violenza, perché deve sconfiggere una violenza superiore. Il suicidio di un giovane precario a vita o di un piccolo imprenditore strozzato da banche senza pietà sono forme di violenza. Certo, una violenza contro se stessi ma pur sempre violenza. Il livello si alza quando la violenza si salda con chi riempie il vuoto dello Stato con la sua subcultura criminale. Come potevate immaginare, signor Ministro, che drammi veri (dalla perdita del lavoro alla diminuzione del potere d'acquisto, dagli indebitamenti all'alea di perdere case e capannoni) non incrociassero la solita strategia criminale di soffiare sul fuoco? Chi doveva tenere sotto controllo questa situazione? Se la sacrosanta protesta di chi viene fregato dal Governo è sporcata dagli scontri, la colpa è del Ministero che non sa proteggere il sacrosanto diritto di dissentire. Ma siccome non volete manifestazioni contro, non avete controllato preventivamente. Le profonde ingiustizie sono sotto gli occhi di tutti e non le voglio elencare: i Benetton che - ahinoi - trattano le migliori condizioni di uscita nella *querelle* sulle concessioni autostradali o Arcuri che non può essere contestato sugli stipendi d'oro perché, nonostante la notizia sia vera, si sente un intoccabile e fa causa ai giornalisti. Insomma, ne abbiamo tantissime. Il problema è che poi ci dite che noi siamo populisti, ma il tema è che i problemi si sono ammalorati nell'incapacità di analisi e di azione di chi avrebbe dovuto avere le leve sotto controllo. Chi pensa di confinare il dissenso e le sacrosante rivendicazioni alla voce «scontri con le Forze dell'ordine» sta facendo male i conti, perché la rete criminale si riprende apertamente la piazza in quanto nessuno l'ha controllata in questi mesi nessuno ha controllato la liquidità messa a disposizione dalle mafie sotto forma di *racket*. Una qualche saldatura tra disperati e criminalità avrà un inevitabile spazio se nessuno blocca, nelle zone più a rischio, lo scivolamento nella disperazione più cupa, fatta di zero lavoro, zero spazi sociali e sloggi dalle abitazioni. Quello spazio di saldatura sarà inevitabile perché, se non si farà vedere lo Stato, si farà vedere l'antistato, il quale agisce *cash* e senza burocrazia. Questa è la grande sfida del Governo. Ministro, il tema di fondo è sempre lo stesso: il controllo del territorio, che abbiamo smesso di fare perché mancano gli uomini e i mezzi e qualcuno ha pensato che, in fin dei conti, ci pensano poi la società liquida e la globalizzazione a rimettere tutto in equilibrio. Non dovete avere paura delle manifestazioni di dissenso; dovete controllare il territorio e proteggere quegli uomini, quelle donne, quei ragazzi e quei giovani che hanno ancora la forza di rivendicare un posto di lavoro e un diritto vero con contratti veri. Dovete aiutare questi ragazzi a poter manifestare senza avere infiltrazioni malavitose.

il Ministro anche per aver sottolineato all'inizio del suo intervento l'impegno del Governo e le cose che ha già fatto per impedire che la criminalità organizzata possa possa avvantaggiarsi della crisi, sfruttandola per favorire l'usura, acquisire locali e costruire consenso sociale. Ministro, prima di tutto le chiedo di esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà agli operatori delle Forze dell'ordine che in questi giorni sono impegnati a difendere le nostre città, ma soprattutto il diritto a manifestare delle persone perbene. Sappiamo che stanno affrontando con misura e attenzione le violenze di piazza, cosa che comporta non solo i rischi consueti ma anche in questa fase il rischio di contagio. Penso, soprattutto nella mia città, al fatto che sono diverse decine gli agenti che si sono infettati con il coronavirus. Signor Presidente, colleghi, c'è nel Paese un disagio evidente e motivato. La ripresa drammatica dei contagi insieme alla crescita delle preoccupazioni per il futuro di fronte alla crisi economica alimentano incertezza e malessere. A ciò si aggiunge in questi giorni l'impatto delle misure che il Governo ha dovuto mettere in campo per combattere la crescita dei contagi senza arrivare al *lockdown*, ma limitando la circolazione delle persone. Queste misure chiedono sacrifici a tutti ma in particolare penalizzano alcune categorie che comprensibilmente hanno protestato, protestano e hanno chiesto ristori al Governo che con il decreto di ieri sono stati garantiti. In questa situazione, soprattutto dove il disagio sociale è più grande, c'è il rischio, che si è già concretizzato, che le giuste preoccupazioni e le fondate paure vengano usate da chi non c'entra nulla con chi legittimamente protesta. Le violenze di questi giorni - lei l'ha detto bene, signor Ministro - non hanno nulla a che fare con le categorie che stanno manifestando in questi giorni. I protagonisti, a seconda delle diverse realtà, sono estremisti violenti, ribellisti, estremisti di destra o di sinistra, frange organizzate nelle curve (c'è il ribellismo); sono le stesse figure legate alla criminalità e alla devianza che spesso incontriamo. Tanti trovano in questa drammatica emergenza l'occasione per sfogare violenza e attaccare le Forze dell'ordine. Di fronte a questa situazione grave ognuno di noi, prima di tutto la politica, ha la responsabilità di intervenire con fermezza, non solo nel contrasto dei violenti ma soprattutto per impedire che la protesta dei violenti si saldi con il disagio sociale. sappiamo, tocca prima di tutto al Governo rispondere e garantire che nessuno sia lasciato solo di fronte alla crisi, interloquire con le parti sociali e le categorie (come ha fatto in questi giorni il Presidente del Consiglio) anche nei momenti più difficili, ma soprattutto dare risposte concrete alle questioni che vengono poste. Lo si è fatto con il decreto di ieri, che garantisce ristori più alti che nel passato a tutte le categorie costrette a chiudere: cassa integrazione e contributi ai lavoratori, dipendenti e non. non basta; serve che quelle risorse arrivino subito e direttamente ai beneficiari. L'impegno assunto di versare direttamente sui conti correnti i contributi entro metà novembre deve essere rispettato;

isolare e prendere le distanze, non mischiarsi con estremisti, violenti e delinquenti. È importante che anche le parti sociali e le associazioni non solo allontanino, ma contrastino i violenti. Ovviamente su questo noi, la politica, abbiamo una responsabilità in più. Sempre, ma ancora di più in una fase così drammatica, la politica deve preservare le istituzioni, la loro credibilità, il loro essere riferimento per tutti i cittadini mentre si sta combattendo un nemico comune che è nemico di tutti. Per questo noi, tutti insieme, abbiamo la responsabilità di rispettare le sedi istituzionali e mantenere i toni giusti in una fase come questa. Siamo tutti impegnati a salvaguardare la salute e l'economia degli italiani. Il problema non è cancellare le differenze o nascondere le contrarietà; ma, più che mai in questo momento, dobbiamo interrompere la campagna elettorale permanente. Il punto non è come si guadagnano o come si perdono i voti, ma assumersi la responsabilità di fare scelte orientate solo a combattere il virus, tutelando salute ed economia. Su questo ci sono opinioni diverse tra noi, ma un Paese ha bisogno di una classe dirigente coesa e unita, capace di condividere l'obiettivo comune di fermare i contagi evitando il *lockdown*. Questo è il modo per isolare e togliere spazio ai violenti: avere grande responsabilità nei toni e nei modi, per essere credibili e avere la fiducia dei cittadini. In un momento in cui più che mai i cittadini hanno bisogno di trovare nelle istituzioni un punto di riferimento rassicurante, serve cercare risposte, non agitare problemi; serve responsabilità. Faccia di più il Governo per coinvolgere in questa direzione tutti, a partire dalle opposizioni. Ma sia chiaro: su questo il Governo può e deve fare di più ma la responsabilità non può stare solo da una parte. Non si può chiedere giustamente di essere coinvolti e poi essere protagonisti delle scene che si sono viste qui ieri, con il capo dell'opposizione che si presenta in Aula e dopo dieci minuti interviene insultando il Governo per poi abbandonare l'Aula insieme a tutto il centrodestra.

Spero si scelga di condividere, ognuno nel proprio ruolo, una parte delle responsabilità, anche per togliere acqua ai violenti e insieme superare, ognuno nel proprio ruolo, questa crisi, questa crisi, non nell'interesse della maggioranza o dell'opposizione ma nell'interesse degli italiani.

non ci sono evidenze di una strategia unica nazionale eversiva e credo che chiunque qui dentro si senta più tranquillo in questo momento dopo le sue dichiarazioni.

in parte anodino, perché ho l'impressione di una Nazione che guarda il dito dell'eversione invece che alla luna del disagio. *(Applausi)*. lo specchio dell'attuale situazione del Paese e credo che chiunque si troverebbe in difficoltà nel guidare il Governo davanti ad una pandemia. È in difficoltà il mondo, ma voi avete scelto una strategia che è discutibile sotto il profilo della legislazione e sotto il profilo degli aspetti costituzionali per l'uso

Siete fermi agli atti amministrativi. *(Applausi)*. La ragione, senatore Mirabelli, per la quale ieri siamo usciti dal Parlamento è perché, nel mentre qui si stava discutendo e il Parlamento stava facendo il suo lavoro legislativo, il Presidente del Consiglio svolgeva una conferenza stampa durante la quale continuava a dire le cose che già l'altro giorno aveva detto in televisione.

e si esercita attraverso una ginnastica e questa ginnastica è la legislazione. La sua salute è la giustizia. Vedo un Governo flebile, debole e noi vogliamo che il Governo sia forte, perché vogliamo che il Paese esca dalla situazione di emergenza. Noi siamo preoccupati e saremo certamente e saremo certamente con il Governo e con le Forze dell'ordine perché non accada e non debba mai accadere che si saldino le difficoltà economiche con coloro i quali vogliono sfruttare gli antagonismi sociali e sovvertire l'ordine democratico, ammesso che vi sia ancora qualche pazzo in questo Paese che pensa a queste cose. *(Applausi)*. Voi allora non ci troverete interessati a cambi di maggioranza o a formule ambigue che non ci interessano. Ci troverete con voi nella misura in cui i vostri provvedimenti sono sostenibili e questo l'ha detto il nostro presidente Berlusconi in modo chiaro e inequivoco. Lo sta dicendo da giorni. Ve lo stiamo dicendo, ma evidentemente siete ancora poco attenti, perché avete paura. Ecco, dovete uscire dalla paura. La paura è una cattiva consigliera e lo si è visto, perché davanti al primo *lockdown* ci siamo trovati impreparati; il Paese lo era, chiunque lo sarebbe stato, lo è stato il mondo. Ma non rispetto a questo ritorno! Rispetto a questo ritorno siamo stati fermi,

se i posti nelle terapie intensive sono stati aumentati oppure no. È mancato il coordinamento dopo la fine della seconda fase. *(Applausi)*. Le Regioni non sempre hanno fatto ciò che avrebbero dovuto. Dov'è l'unità dello Stato tanto invocata, che invocate soltanto a parole nei momenti di bisogno, quando vi serve qualche voto per avere la maggioranza qualificata? Questo è il problema. Il problema è politico. problema. Il problema è politico. Il problema è politico, al punto tale che,

agli eventi appassionanti, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope». Lo diceva Pietro Calamandrei all'Assemblea costituente il 4 marzo 1947. Noi vi chiediamo di saper guardare lontano e ovviamente all'emergenza di questi giorni.

noi rifiutiamo tutti gli atti violenti che si sono succeduti in queste ore nel nostro Paese. *(Applausi)*. Atti violenti che arrivano da forze che fortunatamente non siedono in questo Parlamento e che tuttavia devono essere combattute con determinazione dallo Stato.

bizzarre. Assiste anche lei a una serie di manifestazioni pacifiche: oggi a Roma abbiamo visto almeno quattro manifestazioni pacifiche attorno al Senato e alla Camera dei deputati; tutte manifestazioni pacifiche di cittadini italiani esasperati da questa situazione.

all'altezza del Ponte Regina Margherita, se non sbaglio; il semaforo è diventato verde e ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una guerriglia urbana.

Signor Ministro, e se una di quelle pietre, invece di finire sul porfido fosse finita contro il finestrino di una macchina e avesse creato maggiori danni? Questi sono i problemi che dobbiamo vedere. Signor Ministro, le riporto

Ministro, noi ricordiamo che a marzo in Commissione antimafia già si parlava del rischio di infiltrazioni criminali, quindi già eravate informati di questo rischio. Poi lei ci parla di gruppi di estrema destra, gruppi di estrema sinistra, gruppi organizzati delle tifoserie, e molti di questi si mandano i messaggi sui *social*. Se voi già sapete chi sono e voi lo sapete, perché non posso pensare che uno Stato organizzato non sappia chi sono queste persone perché le Forze di polizia lo sanno - perché non prevenite? Se tutto questo avviene sul *web* e se lei già lo sa, perché non potenziate la Polizia postale, che è quella che dovrebbe controllare queste cose, soprattutto in questi momenti di crisi? *(Applausi)*. Qualcuno diceva che prevenire è meglio che curare. Uno Stato che non prevede e previene gli scontri; l'auspicio è che non vogliate che la situazione sfugga di mano. Vorrei evitare che la situazione sfugga di mano, per poi evitare magari che qualcuno si alzi un giorno e dica: «Visto che le manifestazioni non sono più democratiche, ma sono violente, impediamo agli italiani di manifestare». Voglio evitare che si arrivi a questo livello e quindi magari che ci sia qualcuno che le tolleri per far sì che il livello dello scontro sia sempre più alto. Vorremmo evitare che si arrivi a questo punto. Signor Ministro, secondo me, voi non capite le reali motivazioni che spingono la gente perbene in piazza; non i facinorosi e gli estremisti, ma le persone perbene. Pensate che sia soltanto per i vostri bizzarri provvedimenti? Pensate che sia solamente per la chiusura di alcune attività alle ore 18? No, non è solamente per questo. La domanda è: siete mai andati in piazza ad ascoltare le persone? *(Applausi).* Avete mandato mai qualche vostro parlamentare a dire: «Guardate, sono un parlamentare di maggioranza, vi ascolto e riporto al Governo». Il problema, signor Ministro, è che la gente si sente inascoltata in questo momento. La gente non arriva a fine mese: questo è il problema. Ripeto, la gente che scende in piazza non arriva a fine mese; se lo Stato non l'ascolta, una persona che non arriva a fine mese non sa più che cosa fare se non scendere in piazza a protestare. Il problema grosso è che la gente si sente un numero su cui lo Stato sta facendo esperimenti sociali. Quello che chiedono le persone è reciprocità. I parchi a tema provocano assembramento; gli eventi provocano assembramento; i matrimoni e le cerimonie provocano assembramento; i ristoranti, i bar, i supermercati, i negozi nelle gallerie commerciali, le terme e le palestre: tutto provoca assembramento in questo Paese. E a queste persone si chiede un sacrificio. Bene, queste persone sono anche disponibili a fare un sacrificio, temporaneo, però due cose chiedono allo Stato: innanzitutto, la reciprocità. Cosa vuol dire? Che se un bar provoca assembramento, non posso pensare che un autobus pieno all'ora di punta non sia assembramento. *(Applausi)*. Se una palestra produce assembramento, non posso pensare che un volo di Alitalia sia pieno come una scatola di sardine. Se i ragazzi fuori dalla scuola provocano assembramento, le metropolitane non sono assembramento all'ora di punta? È allora lì che dovete intervenire. *(Applausi)*. Signor Ministro, o tutti o nessuno. La seconda cosa

con le lacrime agli occhi, perché ormai l'azienda è fallita, non può lavorare e deve lasciare a casa 21 persone? *(Applausi).* Gli dite voi che deve andare a casa? Promesse, promesse, promesse!

signor Ministro, il diritto a manifestare le proprie idee, anche quando si è in dissenso con le decisioni delle autorità pubbliche, è sacro e costituzionalmente garantito, ma c'è un altro principio su cui si deve fondare la nostra convivenza civile ed è il rispetto della legalità. In questi giorni abbiamo visto frange di estremisti di destra e di sinistra ed esponenti di gruppi ultras devastare strade e vetrine, saccheggiare e fare tanto altro, da Napoli a Torino, passando per Roma. Ringrazio il signor Ministro per aver detto a chiare lettere che lo Stato intende agire con la massima fermezza contro violenze e strumentalizzazioni, che stanno intossicando il nostro Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pochi giorni fa ha detto una cosa di grande valore, che testimonia la serietà e la consapevolezza con cui lavora il Governo: «Se oggi fossi dall'altra parte, forse anch'io proverei rabbia verso le misure del Governo», perché chi ogni giorno, dalla mattina alla sera, fa i salti mortali per far quadrare i conti, ha anche il diritto di voler sfogare la propria frustrazione. sono però queste le persone che sfasciano le vetrine di Torino, che ribaltano i cassonetti a Roma o lanciano bombe carta a Napoli.

Anche in questi giorni il presidente Conte e altri esponenti del Governo hanno incontrato tanti rappresentanti di queste categorie, si sono confrontati, hanno ascoltato e spiegato. Alla fine prevale sempre la comprensione delle rispettive posizioni e il dialogo accresce la consapevolezza di tutti. I cittadini sanno che un Governo serio e instancabile sta facendo ogni sforzo per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica e sociale. dei ministri è stato approvato solo dopo aver avuto certezze sulle risorse, da inviare in pochi giorni sui conti corrente delle aziende colpite dalle restrizioni, con importi pari o superiori ai trasferimenti a fondo perduto, decisi con il decreto rilancio. Stiamo facendo il massimo, in un contesto da far tremare le vene ai polsi di qualsiasi statista: è sufficiente vedere cosa succede al di là delle Alpi. non si può dire lo stesso per qualche esponente delle opposizioni che, dopo mesi di chiacchiere a vuoto, speculazioni vergognose su una tragica pandemia, tra negazionismo e allarmismo alternati ad arte, in base a dove gira il vento, ha definito «cretini» i manifestanti violenti di questi giorni. Il senatore Salvini - che non vedo in Aula stasera - di parole forti ne ha usate tante. Dovrebbe prendere le distanze, invece, da frange di delinquenti. Questo è il termine corretto: «delinquenti» che inquinano la democrazia, colpiscono al cuore lo Stato di diritto e sfruttano in modo ignobile rabbia e sofferenza di lavoratori perbene. Abbiamo a che fare con criminali, a cui lo Stato non deve fare sconti in nome della dignità e della serietà di ogni cittadino perbene. Anzi, lo Stato dovrebbe prevenire ed evitare che dilaghi la paura. Nessuno si tiri indietro dal dire, ad esempio, che una formazione politica notoriamente estremista e violenta come Forza Nuova ha messo a ferro e fuoco il centro storico di Roma. Le loro scorribande non hanno nulla a che fare con la libertà di manifestare, perché chi compie simili violenze si colloca sempre dalla parte del torto. Si può prevenire. Tutti noi dentro quest'Aula, per parte nostra, abbiamo il dovere di farci carico e sentire come un'angoscia personale la sofferenza di chi, esasperato da una situazione inimmaginabile appena un anno fa, sfoga tutto il proprio disappunto e le proprie preoccupazioni in piazza. Per fortuna, l'Italia si è trovata ad affrontare una tempesta senza precedenti con un Governo responsabile e che lavora. *(Applausi).* L'attività legislativa e amministrativa messa in campo in questi mesi è paragonabile al lavoro di anni e anni. Adesso bisogna compiere ogni sforzo affinché a nessuno sia più permesso di agire al di fuori della legalità. Prima di concludere il mio intervento, mi sia permesso un sincero e profondo ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine *(Applausi)*: padri, madri, fratelli e sorelle di famiglia, che con serietà e professionalità difendono la nostra sicurezza in questi giorni così difficili. Questi sono i coraggiosi cittadini a cui cittadini italiani guardano con fiducia. La nostra democrazia forte non si farà impressionare da una bomba carta o da un cassonetto incendiato.

che, contrariamente ad alcuni colleghi, sono pienamente soddisfatto di quello che il Ministro ha detto. Noi non l'abbiamo chiamata per fare lezioni di sociologia né per spiegare quello che sappiamo benissimo - perché sarebbe insultante prima di tutto verso di noi, se avessimo bisogno che qualcuno ce lo spieghi - e, cioè, che c'è uno stato di disagio profondo e di protesta forte nel Paese. Aggiungo, da persona che vota questo Governo, che tale protesta è pienamente legittimata perché, purtroppo, in una pandemia di questo tipo, chi perde il lavoro o chi deve chiudere le sue attività commerciali è ovvio che sia profondamente frustrato. Non avevamo bisogno del Ministro dell'interno per capire questo. Abbiamo quei minimi contatti sociali, nonostante il distanziamento sociale, che ci portano a dire che lo avevamo immaginato anche da soli. Il Ministro dell'interno è stato chiamato per parlare di quello che è successo in questi giorni, che nulla ha a che fare - come ha detto poc'anzi la collega - con la giusta, legittima (e da tutelare) protesta che c'è nel Paese. Anzi, è proprio la garanzia di questa protesta civile che dobbiamo alzare le barriere contro quel misto e quell'impasto di violenza, di delinquenza, di camorra, di centri sociali, di estremisti di destra che si stanno muovendo in questo momento e che si stanno muovendo nelle città che sono state bersaglio degli scontri. Il Ministro si è attenuto a questi fatti ed è giusto che lo abbia fatto, perché io ritengo assolutamente sbagliato che noi mischiamo questo stato di disagio, che esiste e che può avere anche giustificazioni di qualsiasi tipo, con quello che invece non è giustificabile.

il destino comune di questo Paese. Vorrei ricordare a loro che durante l'epoca del terrorismo, nonostante ci fossero circoli intellettuali che teorizzavano né con lo Stato né con le Brigate Rosse, ci fu qualcuno, ed era allora all'opposizione dei Governi guidati dalla Democrazia Cristiana, che non ebbe incertezze e si schierò per lo Stato democratico contro i violenti. Se le istituzioni hanno retto e se anche chi allora era all'opposizione ha maturato negli anni una legittimazione istituzionale, è stato perché in queste circostanze ha saputo scegliere la parte in cui collocarsi. collocarsi. Amici, anch'io ho molte cose da dire, le dico ogni volta che viene il Presidente del Consiglio: mi piacerebbe una maggiore assertività del Presidente del Consiglio nel coinvolgere l'opposizione; non mi piace che l'opposizione sia consultata cinque minuti prima con una telefonata, perché questa è una consultazione retorica. Mi piacerebbe che ci fosse la convinzione che dobbiamo andare avanti assieme; il senatore Mirabelli ha detto delle cose che condivido dalla A alla Z e anche il collega Dal Mas credo abbia manifestato una sensibilità che esiste;

abbia biasimato il Presidente del Consiglio perché in quel momento parlava alla televisione mentre erano in corso i lavori parlamentari; su questo non dico se ha ragione o torto, probabilmente ha anche delle motivazioni, poi ha chiesto all'opposizione di abbandonare l'Aula e se ne è andato via. Guardate che non funziona così! *(Applausi)*. Se c'è qualcosa da biasimare nei confronti della maggioranza e si sta dentro al Parlamento e lo si rileva in Parlamento, forse si ha maggiore legittimità per dire che il Presidente del Consiglio sbaglia, altrimenti si finisce per dare l'idea che si vuole solamente cercare un pretesto per fare l'ennesima polemica con la maggioranza.

ma con la capacità, ognuno nel suo ruolo, di essere responsabili, di capire che il momento ci chiede un'assunzione di responsabilità. E il ministro dell'interno dell'interno Lamorgese deve andare via questa sera sapendo che lei, la Polizia, i Carabinieri le Forze dell'ordine hanno la solidarietà di tutto il Parlamento, che non ci sono dei distinguo. *(Applausi)*. Non mi piace che si dica: il Ministro ha ragione, però. No, colleghi, il «però» non esiste. Il Ministro ha detto le cose come stanno e ha detto che lo Stato non si farà intimidire dai violenti e dai delinquenti e su questo deve poter contare su tutti noi, su chi sta nella maggioranza e chi sta all'opposizione. Per me il senso di questa comunicazione è esattamente questo e la mia solidarietà è senza condizioni.

vetrine infrante, lanci di bottiglie incendiarie contro la Polizia, cassonetti dei rifiuti messi a fuoco, negozi derubati: sono le scene di guerriglia urbana che hanno caratterizzato le ultime 48 ore praticamente su tutto il territorio nazionale, ieri sera anche a Roma. Le proteste contro il decreto Covid, prima pacifiche, sono poi diventate un'altra cosa. Si sono trasformate in violenza attraverso l'infiltrazione di gruppi di estrema destra, di movimenti antagonisti di *ultras*, di esponenti del crimine organizzato, che provano a cavalcare la tensione di queste ore e diventare interlocutori della protesta aizzandola. A Piazza del Popolo, ieri sera, non c'erano solo i *leader* di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, a fagocitare le cariche e a tirare transenne contro la Polizia e i Carabinieri, ma c'erano numerosi loro militanti, professionisti della violenza, che si insinuano nelle proteste e le alimentano per strumentalizzare e provocare disordini a Roma come nelle altre città, dove si è manifestata una pericolosa commistione, quindi, tra estremisti delle destre neofasciste e appunto altre varie frange, in alcuni territori anche esponenti della criminalità organizzata, tutti soggetti con una forte propensione alla violenza che aizzano e danno sfogo alla rabbia che sta montando nel Paese; tutti soggetti che vanno individuati e perseguiti in modo esemplare, perché non è ammissibile che si approfitti di situazioni di difficoltà come quella in corso per indurre chi è esasperato a commettere a sua volta atti di vandalismo. Al contempo, il nostro grazie più sentito va alle Forze dell'ordine ed è positivo che sia un grazie *bipartisan*, non solo da parte del nostro Gruppo, perché non è accettabile tollerare le forme di violenza a cui abbiamo assistito nelle ore scorse. Ecco perché, signor Ministro, riteniamo che oltre ad individuare i responsabili, oltre ad esprimere la nostra solidarietà alle Forze dell'ordine, sia giunta l'ora di applicare la legge Mancino e procedere con lo scioglimento di Forza Nuova, un'organizzazione che persegue un'ideologia neofascista, che ha più volte causato violenti scontri con la Polizia, che è autrice di ripetute intimidazioni nei confronti di singoli esponenti politici e che anche in queste ore aizza appunto all'odio in diverse piazze italiane. Persegue un disegno criminale di inquinamento e proprio per questo è necessario che lo Stato intervenga con decisione e senza tentennamenti ed è giusto il suo richiamo, signor Ministro, a non lasciarsi strumentalizzare e a prendere invece le distanze da tali provocatori. Allo stesso tempo, signor Ministro, è necessario avere presente che tra chi è sceso in piazza in questi giorni non ci sono solo facinorosi, non ci sono solo criminali, c'è anche una moltitudine di gente per bene che esprime la propria disperazione, scendendo in piazza vuole dare voce alla propria angoscia, alla paura di vedere andare in fumo la propria esistenza professionale a causa delle chiusure decise dall'ultimo Sono ristoratori, proprietari di bar, titolari di cinema, ambulanti, gestori di centri sportivi, piccoli imprenditori, che nelle scorse settimane hanno fatto investimenti consistenti, si sono attenuti alle regole, hanno fatto di tutto per garantire condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal Governo per sanificare i locali, per distanziare i clienti, gente che adesso, dopo aver subito forti cali negli incassi e dopo aver fatto grossi sacrifici, pur di tirare avanti, si vede minacciata nella propria sopravvivenza economica. Sono imprenditori che chiedono di poter lavorare in sicurezza per sé e per i propri dipendenti, nel totale rispetto delle regole, per la salvaguardia della salute propria e dei rispettivi clienti, perché anche se forniremo loro uno, due o tre mesi di sussidi, sanno che prima o poi questi aiuti finiranno e per quanto essenziali gli importi non saranno sufficienti per la loro riapertura. Il tutto a seguito di un decreto - diciamocelo - che rischia di più di essere basato su delle suggestioni che non su dati scientifici e mentre è assodato che purtroppo le scelte assunte bloccheranno determinati settori dell'economia, è del tutto da verificare che saranno altrettanto efficaci nel bloccare il numero dei contagi. Allora, signor Ministro, così come siamo convinti che le regole vadano rispettate e che i violenti vadano puniti, allo stesso modo crediamo che sia necessario ascoltare la voce dei tanti cittadini onesti scesi in piazza in modo pacifico in queste ore, così come riteniamo che vadano ascoltate le voci delle opposizioni e anche di chi, all'interno della maggioranza, usa toni critici ma non certo

a nome di Fratelli d'Italia, per la galanteria e il rispetto che caratterizza il nostro partito,

Abbiamo ascoltato con attenzione le sue parole, però ci poniamo una domanda. Ce la siamo posti, per la verità, già ieri quando abbiamo sentito il Partito Democratico chiedere il suo intervento.

sul quale il Parlamento non ha avuto modo di dire una parola, sarebbe stato nettamente più conveniente e opportuno, per il rispetto delle istituzioni democratiche, che in questo Senato fosse presente il Presidente del Consiglio dei ministri. Amici del Partito Democratico, capiamo

scomodare il Ministro dell'interno e sentirsi dire che sono avvenuti degli scontri di piazza, ma che fondamentalmente le Forze dell'ordine, correttamente con tutto il nostro supporto, hanno fatto il loro dovere.

ministri ha spaccato il Paese per davvero. Siete riusciti a dividere gli italiani; siete riusciti a dividere gli operatori economici del nostro Paese e questa è una cosa molto grave. Vorremmo capire da parte

sono ossequienti e obbedienti e il giorno dopo si svegliano per fare l'opposizione nella maggioranza o se, invece, come ha risposto Rosato, sono le osservazioni non ascoltate del giorno prima. Queste sono la maggioranza e la sua dialettica, che è più che altro

a nome di Fratelli d'Italia, un no chiaro e deciso a ogni forma di violenza. Esprimiamo la più grande solidarietà ai valorosi militi, ai carabinieri, ai poliziotti e alle Forze dell'ordine, che purtroppo sono lasciati, anche per colpa vostra, allo sbaraglio di fronte a questa situazione. Tra l'altro, sono spesso privi di attrezzatura e con stipendi non certo all'altezza del ruolo che svolgono nell'interesse di tutti noi.

ha tutto il diritto di poterlo fare. Noi di Fratelli d'Italia siamo e saremo sempre al fianco dei nostri lavoratori, degli imprenditori, dei commercianti, dei ristoratori, dei titolari delle palestre, di tutti coloro che voi

Sono trascorsi otto mesi, più o meno, da quando è scoppiata la pandemia. Avevate tutto il tempo per investire quel denaro, che oggi volete investire a debito del nostro Paese, nella giusta assistenza: perché, a questo punto, diventa una giusta e doverosa assistenza. Quel denaro, però, avreste potuto investirlo nella prevenzione, in modo tale da non trovarvi, oggi, nella condizione di dover chiudere il Paese. Se penso voi cosa avete fatto? Cosa avete fatto per risolvere uno dei maggiori problemi che ruota intorno alla pandemia e alla diffusione del virus, cioè il trasporto pubblico? Non avete fatto nulla! Voi ritenete che siano più pericolose le palestre, dove hanno attuato investimenti e dove le macchine per fare sport distano metri l'una dall'altra, piuttosto che gli assembramenti nelle metropolitane o sulle corriere. Ecco perché vi accuso, a ragion veduta, e vi accusano gli italiani di incapacità, di non aver saputo interpretare i bisogni del nostro Paese, i bisogni di quei lavoratori che voi avete trascurato e che oggi, semplicemente aumentando il debito degli italiani, dite di essere pronti a ristorare: peraltro malamente, come poi dirò. ministri, d'altra parte, è figlio di quel pauperismo e di quella visione etica che contraddistingue, purtroppo, la vostra maggioranza politica, la vostra visione politica di sinistra, quasi consona e affine a quella teologia della liberazione per la quale, magari, si può andare giustamente in chiesa, ma non si può andare in palestra, non si può andare al ristorante, perché quelle attività sono, come qualcuno di voi ha detto, superflue.

Quindi, ristoro e nuovo debito per venir meno agli investimenti che non avete saputo fare. Trasporti, servizi sanitari, assistenza domiciliare agli anziani, scuola: non avete fatto nulla in sei mesi, tranne i monopattini, da una parte, e banchi a rotelle, dall'altra. Adesso, allora, dovete coprirvi alle spalle degli italiani e dovrete indebitare ancora di più il Paese per coprire le vostre inefficienze. Lo dico e lo ripeteremo a voce alta dappertutto: nelle città, nei paesi, nei rioni della nostra amata Patria. Ebbene, parlate anche di ristoro e qui dimostrate l'incompetenza aziendale del vostro agire. Ma come pensate di ristorare gli italiani con l'elemosina? Voi avete detto e scritto che il ristoro sarà comparato a quello del decreto di giugno. Allora, il decreto citato prevede un contributo a fondo perduto che varia dal 10 al 20 per cento sulla riduzione dei ricavi. Cosa vuol dire, tradotto in poche parole? Che voi forse a malapena ristorerete una parte dell'utile di queste imprese. Ma i costi fissi che queste imprese devono comunque sopportare chi li paga? Li pagate voi? allora, il coraggio di essere più onesti intellettualmente. Abbiate il coraggio di ascoltare chi sta urlando e protestando nelle strade. Altro che parlare dei violenti. I violenti vanno repressi e mi auguro che il Ministro dell'interno sappia svolgere le sue funzioni a tal riguardo. Chi protesta ha il dovere e il diritto di farlo, perché voi li state ignorando. E anche quando parlate di ristoro, li state prendendo in giro, perché ribadisco che con il 10, 15 o 20 per cento del minor fatturato non si ristora un bel nulla, ma - semplicemente - si spendono

che spero vorrà risponderci con chiarezza, che provvedimenti ha preso verso quegli immigrati clandestini che continuano a invadere il nostro Paese e scappano dai centri, magari malati di Covid. Che provvedimenti state prendendo verso gli immigrati clandestini? Lo vorremmo sapere, visto che volete chiudere in casa gli italiani e impedire ai nostri ristoratori di lavorare, dopo che magari - faccio una parentesi - hanno investito fior di soldi per garantire il distanziamento e la sanificazione. Dopo che hanno investito soldi, li fate chiudere! Impedite anche che le famiglie possano festeggiare il compleanno di un figlio, però,

Non vorremmo che questi disordini e magari le violenze che, ahimè, spesso si accompagnano alla disperazione sociale sociale vi facessero comodo, perché è attraverso questi elementi che voi potrete conservare il potere. Volete solamente la poltrona; è la poltrona che vi interessa e non certo il destino e le sorti della nostra Patria.

Signor Ministro, abbiamo tutti ascoltato con attenzione e preoccupazione la sua informativa. Le chiedo anche io, a nome delle colleghe e dei colleghi del Gruppo Misto, di esprimere la nostra solidarietà alle Forze dell'ordine aggredite nel corso delle manifestazioni violente di questi ultimi giorni. *(Applausi)*. Signor Ministro, questa è l'ora più buia per il nostro Paese dal Dopoguerra. Quella che, alla fine dello scorso febbraio, si era palesata come un'emergenza sanitaria è diventata rapidamente e drammaticamente anche un'emergenza economica e sociale, che in questa seconda ondata sta mettendo a dura prova la coesione sociale e rischia di mettere in discussione la tenuta democratica del nostro Paese. Oggi dobbiamo fare i conti con due emergenze contemporaneamente: quella sanitaria e quella economica. Giorno dopo giorno si riempiono di nuovo gli ospedali e le terapie intensive, aumenta il numero dei morti, il contagio corre veloce (solo oggi 25.000

delle attività del terziario e della ristorazione, necessarie per ridurre il contagio, hanno portato in piazza, colpiti dalla crisi economica, ceto medio, piccola borghesia e marginalità e, con loro, gli ultimi degli ultimi: precari, disoccupati e addetti di quel sommerso che alimenta anche la criminalità, ma che non è solo funzionale alla criminalità, in quanto fa sopravvivere migliaia di persone, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Piazze composite con diversi protagonisti, quei ceti impoveriti dalla pandemia e i protagonisti di quelle immense periferie che sono diventate le nostre metropoli; piazze esposte all'egemonia della destra, del tutti contro tutti, del rancore, dell'invidia sociale e del ribellismo. In queste piazze abbiamo sentito gridare contro la dittatura sanitaria, contro lo Stato. Per loro il nemico da abbattere non è il virus, ma i provvedimenti presi per contrastarlo; su queste proteste si innesta di tutto. Signor Ministro, colleghe, colleghi, la gente è spaventata, disorientata. È un momento in cui c'è tanta sofferenza e in cui migliaia di persone si sono trovate senza lavoro. Saremmo tutti più tranquilli se dietro a queste manifestazioni avessimo individuato un'unica regia criminale. Certo, è vero che negli scontri di venerdì sera a Napoli, sotto la Regione Campania, c'erano i malavitosi, gli ultrà, gli antagonisti di sinistra e il giorno dopo, nel quartiere del Vomero, quelli di CasaPound, che hanno tentato di egemonizzare la protesta; come erano di Forza Nuova i manifestanti che hanno provocato gli scontri di ieri a Roma a Piazza del Popolo. Ecco, dobbiamo chiedere a chi legittimamente manifesta nelle strade delle nostre città di isolare i violenti e di rispettare le regole. Sappiamo che magistrati e investigatori sono al lavoro per identificare gli autori di queste violenze; ci sono forze criminali ed eversive che soffiano sulla protesta. Ma, attenzione, in queste piazze non c'era solo rabbia; c'era paura, paura per il futuro,

per quelle attività chiuse di sera. Bene ha fatto il Governo a prolungare di altre sei settimane la cassa integrazione e a estendere lo stop ai licenziamenti. Bisogna pensare a sostenere economicamente anche gli invisibili; occorrono risposte concrete. Abbiamo già chiesto a marzo e ad aprile sforzi al limite dell'impossibile alla nostra comunità e lo stiamo facendo ancora, a distanza di otto mesi; e sarà così ancora nei mesi a venire. Dobbiamo continuare a tenere dritta la barra e a mettere al primo posto il diritto alla salute. Non siamo i soli a soffrire per gli effetti della pandemia; non dimentichiamoci mai quello che sta accadendo in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, nel resto del mondo. Dalla sua informativa, signor Ministro, si capisce bene che lei e il Governo non sottovalutate la situazione; è legittimo protestare anche in tempi di emergenza sanitaria, con le regole, però, che questa emergenza impone. Voglio chiudere questo intervento rivolgendomi a quest'Aula: non è il momento di cavalcare le proteste, non è il momento della propaganda. Ognuno si assuma le sue responsabilità: maggioranza e opposizione. Abbiamo il dovere di confrontarci, per combattere il Covid e per rispondere alla crisi economica e sociale. Signor Ministro, noi siamo d'accordo con lei: bisogna essere fermi e rigorosi nel bloccare odiatori ed eversori. Dobbiamo invece spendere tutto il nostro impegno nel rispondere al disagio sociale con politiche che riducano le diseguaglianze. La posta in gioco è il futuro del nostro Paese, anzi del nostro pianeta.

ho ascoltato con molto interesse la relazione del Ministro dell'interno, perché ci ha riportato alla logica dei numeri - e qui non si può scherzare rispetto a dare l'idea che il Paese ha delle piazze che bruciano, spostando l'attenzione su quello, quando invece sappiamo che il tema è l'emergenza sanitaria e la la salute e la dignità delle persone e il diritto al lavoro e all'educazione dei nostri figli. Quindi bene che abbia dato la giusta contezza dei numeri, perché dobbiamo partire da lì e non dall'emotività, non dalla strumentalizzazione politica, pur sapendo che oggi siamo in una fase nuova, che è cambiata anche rispetto a marzo e ad aprile, quando era naturale abbracciarsi e unirsi intorno alle autorità precostituite. Oggi è più complicato, perché non c'è più l'incognito. Oggi il virus lo conosciamo, conosciamo le sue dinamiche, o almeno la maggior parte di esse, seppur differenti da territorio a territorio. Vivo in Lombardia: tra Milano e Varese le ultime notizie danno un aumento di oltre 7.500 casi; nella mia provincia, quella di Varese, quasi 2.000 casi nella sola giornata di è differente tra settore e settore, perché chi lavora nel pubblico e fa lo *smart working* ha evidentemente una sensazione e una percezione diverse rispetto a chi lavora nel settore privato, ad esempio quello dei ristoranti e dei bar. Quindi, comprendiamo la preoccupazione ed è fisiologico che molte persone vogliano manifestare la propria preoccupazione sul futuro, le proprie ansie e inquietudini, e noi dobbiamo farcene carico. Volevo dire in maniera molto chiara a chi è stato Ministro, come il senatore

Puoi avere vedute diverse rispetto a quelle del Governo, così come il sindaco di un'importante città italiana che, ieri, alle ore 5 del mattino, non ha trovato altro da fare che andare a cena con altre persone nello spregio più totale delle norme di distanziamento. Chi ha un incarico istituzionale deve dare l'esempio; poi può discutere sulle singole misure, arrabbiarsi, dividersi, ma non possiamo permetterci di mettere in discussione il principio di legalità. Ci riempiamo molto spesso la bocca della parola «legalità», ma dobbiamo poi essere conseguenti. essere attenti ed è bene che tutti condannino "senza se e senza ma" gli episodi di violenza, senza sponde istituzionali, perché ormai con i *social* e i mezzi di comunicazione le persone si nutrono di messaggi sbagliati. E, se si pensa che qui dentro qualcuno dà la sponda sul versante dell'illegalità e del non rispetto delle regole, si dà spazio a persone che invece si muovono per tutt'altro. Occorre distinguere tra chi giustamente è preoccupato per il futuro, che va compreso, e chi invece scende in piazza per motivi diversi: dall'antagonismo ai movimenti neofascisti, dalle bande giovanili delle curve che sono in contatto con i delinquenti in servizio permanente effettivo. Vorrei provare a fare un richiamo che riguarda tutti, a livello locale come a livello nazionale: il momento della responsabilità collettiva vale per tutti. Significa che chi fa parte della classe dirigente del Paese deve cambiare modo di rapportarsi rispetto a questa crisi, a partire da noi, a partire da chi è forza di maggioranza a partire dagli stessi sindacati, dalle forze sociali alle associazioni di categoria. Bisogna essere consapevoli che oggi non si è solo portatori di un interesse di parte, ma si è anche componente effettiva della classe dirigente del Paese e, quindi, va cambiato l'atteggiamento nei confronti della crisi: vale anche per le forze di maggioranza, che giustamente devono essere coinvolte anche con modalità innovative, a partire dalla funzione di raccordo dei Capigruppo che tengono il collegamento fra Governo, Gruppi e territorio. Si discuta dentro quel formato nuovo, poi si decide, magari mediando, magari con discussioni accese, ma poi quando si esce non si giocano altre partite, perché non ce lo possiamo permettere. La partita oggi è affrontare insieme il Covid-19. Quindi, lasciamo stare i regolamenti di conti e pensiamo a come affrontare insieme l'emergenza e vale per le forze di opposizione che chiedono giustamente un coinvolgimento non di cortesia. Però decidiamoci, perché stridono le parole di oggi di un uomo di Stato - voglio dirlo - qual è Silvio Berlusconi rispetto alle sceneggiate che abbiamo visto qui ieri di chi ha abbandonato l'Aula, perché si rimane in Aula e si svolge il proprio ruolo. Questo è un punto fondamentale che riguarda anche il centrodestra. Dovete decidere che cosa fare:

velocità e condivisione delle scelte. Se dobbiamo affrontare questa sfida, dobbiamo mettere in campo strumenti anche nuovi. Vale per la cabina di regia, vale per il coinvolgimento dei Capigruppo: decidiamo quali sono le modalità. E vale anche - lo dico al Ministro dell'interno - rispetto alle modalità di organizzazione sul territorio: i prefetti operano ancora con il formato del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica o si inventano formule nuove di *governance* del territorio, cui

Non è che, se perde il Presidente del Consiglio, poi vince il resto del Paese. Oggi ognuno si prenda la propria parte di responsabilità, a seconda dei ruoli e degli incarichi che ha, e risponderà per questo al Paese.

Ministro per la solerzia con la quale ha voluto intervenire questa sera, dandoci delle assicurazioni. Ci ha detto che non saranno limitati i diritti dei cittadini di manifestare democraticamente e di rappresentare le critiche ai provvedimenti del Governo; ci ha detto che saranno isolati, individuati e assicurati alla giustizia i fomentatori, gli estremisti, i provocatori che si insinuano nel malessere dei cittadini per altre finalità.

Qualche mese fa circolava un documento, che non è stato mai smentito - anzi è stato confermato - datato gennaio 2020, nel quale si diceva che la pandemia sarebbe durata moltissimi mesi e avrebbe provocato circa 50.000 decessi. Questo documento non soltanto non è stato smentito, ma è stato anche confermato. Alla legittima domanda di chi ragione questi dati fossero stati tenuti riservati, è stato risposto che era stata una scelta politica per evitare allarmismi. Molto bene, se se questo però avesse significato per il Governo adottare tutte quelle iniziative e tutti quei provvedimenti che avrebbero consentito di affrontare l'emergenza. Signor Ministro, con il *lockdown* di qualche mese fa si è data l'impressione che sarebbe bastato poco più di un mese di privazione forzata della libertà e dei movimenti per debellare la pandemia. E, invece, l'abbiamo mandata soltanto in ferie, perché dopo l'estate l'abbiamo rivista ancora più agguerrita e ancora più violenta di prima. Questo manifesta un'assoluta mancanza di programmazione e una incapacità di affrontare le problematiche. Oggi siamo costretti a prendere atto di iniziative violente di pochi facinorosi che si mobilitano e si inseriscono in certi contesti. Anche io, signor Ministro, voglio manifestare per il mio Gruppo la vicinanza, la stima e la considerazione a tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine. Tuttavia - e qui c'è la differenza - mi consenta, a titolo personale, di esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà a quel poliziotto che a Parma è stato sospeso mentre svolgeva il proprio dovere e mentre evitava che un facinoroso colpisse la vetrina di un negozio, aggredendo la proprietà privata, che ancora nel nostro Paese è garantita. *(Applausi)*. In questa maniera si mostrano solidarietà e vicinanza alle Forze dell'ordine. come esponente parlamentare, ma anche come figlio di una famiglia di tutori dell'ordine che ha visto le frustrazioni e le mortificazioni degli appartenenti alle Forze di polizia, e ha vissuto le ansie, i dolori, le pene e le sofferenze delle famiglie. Allora basta con le parole di occasione: manifestiamo concretamente la vicinanza alle Forze di polizia e incominciamo ad adeguare gli stipendi, che sono i più bassi d'Europa.

per tornare alla situazione precedente, che già non era rosea. Il Governo non ci dice niente su come affrontare la situazione. In Germania, al primo apparire della pandemia, sono stati stanziati 500 miliardi di euro; in America 1.000 miliardi di dollari; da noi, dopo nove mesi, poco più di 100 miliardi, e non tutti sono arrivati a destinazione! Voi pensate in questa maniera di poter affrontare la situazione? tutti insieme dobbiamo fronteggiarla. Signor Ministro, deve dire al Presidente del Consiglio che noi leggiamo dichiarazioni di disponibilità da parte del segretario Zingaretti, da parte del presidente Renzi, ed oggi le abbiamo sentite anche dal presidente Casini che, peraltro, già in altre occasioni le aveva manifestate. Ma nei fatti questo non c'è, nei fatti questo non c'è, perché «collaborare» e «disponibilità» significano decidere insieme in un momento delicato nel quale è in discussione non la sorte di questo Governo, che ci interessa ben poco, ma la sorte e la vita del nostro Paese.

Allora, a chi si è risentito del gesto compiuto ieri dall'opposizione, voglio dire che in questi mesi sui tantissimi vostri decreti-legge, peraltro subiti con il voto di fiducia - quando abbiamo potuto discuterli, perché più il più delle volte li abbiamo ricevuti e dovuti votare così come sono arrivati dalla Camera dei deputati - non si sono accettati gli emendamenti. Non esiste più l'ostruzionismo parlamentare: è stato abolito. Non si fanno più le manifestazioni e non si coinvolge l'opposizione. Che cosa deve fare l'opposizione per dire che prende le distanze da questo modo di fare politica *(Applausi)*, se non abbandonare l'Aula in segno di protesta per attirare l'attenzione dei cittadini, ma anche per sensibilizzare il Presidente del Consiglio e le forze di Governo? È all'interno delle forze di questa maggioranza che esiste il problema.

e convochi le opposizioni, che saranno in grado di assumersi le loro responsabilità *(Applausi)* e anche di dare dei buoni consigli.

che non basta dire che noi affrontiamo i nostri problemi se poi in questi mesi non si sono aperti gli ospedali che erano stati chiusi per poter fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Se ci sarà la chiamata dell'opposizione, come sempre, con senso di responsabilità, noi diremo: presenti.

Signor Ministro, inizierò con una riflessione che ho fatto prima, quando entrando ci siamo stretti la mano, in maniera assolutamente corretta, e lei, con una battuta quasi scherzosa, ha detto: «Ecco il mio nemico». Non è questo lo spirito con cui ci vogliamo rapportare con il Governo, riguarda lo spirito non tra due persone che si conoscono, ma tra le istituzioni. Noi rappresentiamo, in Parlamento, l'opposizione. Vogliamo chiamarla minoranza? Chiamiamola minoranza. Dall'altra parte, infatti, c'è non il Governo, ma la maggioranza. Ciò che stiamo cercando di dire è che quelle che portiamo in questa sede non sono angosce campate in aria, ma sono le preoccupazioni di un Paese che è in grave crisi, innanzitutto le rassicurazioni che oggi avremmo voluto sentire da lei, sono quelle che deve dare il Ministro dell'interno, allorquando in piazza scendono cittadini, che hanno legittime aspettative e gravi preoccupazioni sul loro futuro *(Applausi)*, ma che si trovano mescolati

ebbe l'attenzione di sottolineare i rischi l'11 luglio, ma è evidente che la sua voce è rimasta inascoltata da parte di tutto il Governo, perché le condizioni in cui ci troviamo oggi erano ampiamente

mescolato assieme a chi le regole le calpesta sistematicamente, perché è criminale. Lo dico alla senatrice Mantovani, che non vedo in Aula, perché alle ore 18 se n'è andata: noi abbiamo preso posizione subito.

Non sono questi i toni che si possono usare in quest'Aula, chiedendo poi collaborazione all'opposizione, perché quella battuta scherzosa, fatta tra di noi prima, qualcuno la sta interpretando sul serio, pensando che da questa parte non ci sia qualcuno con cui collaborare, ma c'è il nemico.

sono distanti dai cittadini, dagli operatori economici, dai commercianti e dagli artigiani. E - vivaddio! - non andiamo a dire che sono loro che devono prendere le distanze dai facinorosi! Signor Ministro, c'è qualcosa che è scappato anche in un'intervista.

Le chiedo anche di precisare il suo pensiero, perché nel Resoconto stenografico, che è stato pubblicato nella pagina Internet del Senato, viene riportato che lei avrebbe detto, poco fa - a me è sfuggito, ma le chiedo di precisarlo era presente in piazza un gruppo di 400 persone, a Milano, «tra cui appartenenti all'area anarco-antagonista milanese e un folto gruppo di giovani, nonché soggetti del mondo del lavoro autonomo», che ha provocato vari danni. Dubito che si riferisse al mondo autonomo perché, se si va a dire che in piazza c'erano dei facinorosi geometri, architetti e professionisti, veramente si arriva al paradosso. Ministro, siamo preoccupati perché queste sono le informazioni che vengono pubblicate dai giornali: arrestati due pregiudicati a Napoli e già scarcerati, liberi. State varando decreti. Prendete provvedimenti perché questi fatti non accadono. Se ci sono facinorosi che vanno in piazza, devono essere arrestati e carcerati e non liberati, altrimenti abbiamo un'altra preoccupazione, Ministro. Ci ricordiamo di questa primavera, quando nelle carceri ci furono sommosse: l'*affaire* Basentini, ricordiamo bene che cosa accadde; le pressioni che in seguito furono descritte come fatte sul Governo per liberare e scarcerare. Non vogliamo immaginare che in questo momento ci sia un'idea di infiammare le piazze per fare pressione sulle istituzioni repubblicane per trarne vantaggio da parte della criminalità organizzata, che sia mafia, camorra o 'ndrangheta, perché questo necessiterebbe della massima determinazione nella repressione. E questa massima determinazione nella repressione la chiediamo e pretendiamo dal Governo, distinguendo i cittadini perbene dai facinorosi, e garantendo, ai cittadini che hanno necessità di manifestare tutta la loro situazione, la libertà di farlo in una piazza non violenta. Ministro, abbiamo bisogno di queste certezze. Esistono anche i Servizi nel nostro Paese, che evidentemente fanno il loro dovere, ma mi viene da dire: è possibile che si fossero formate quelle aggregazioni nelle piazze, mescolando come è scritto nelle informative della DIA - camorristi? Non è possibile, non è ammissibile che avvenga, quando lei stessa l'11 luglio disse di fare attenzione perché il rischio c'era, e forte. Dopo di me interverrà il senatore Morra, che sicuramente ci farà un'ampia illustrazione dell'attività di malavita-criminalità organizzata, ma noi vogliamo sentirlo da lei, Ministro. Vogliamo avere la certezza che le nostre istituzioni stanno lavorando per rassicurare i cittadini, e non per dire loro di non andare in piazza perché è pericoloso, ovvero mettere un bavaglio a chi in questo momento si è visto chiusa l'attività, a chi in questo momento non capisce perché gli sono state imposte regole ingiuste. Noi siamo qui per dirvi - come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto - di non prendere decisioni dalle quali il Paese può uscire drammaticamente sconvolto. Avete messo delle regole, Avete messo delle regole, la distanza, regole di buonsenso: fatele applicare, altrimenti far chiudere tutto vuol dire che il Governo fa norme che poi non è in grado di applicare, e chi le ha rispettate si trova addirittura ad essere "cornuto e mazziato". Questo non è ammissibile. vogliamo rassicurazioni certe per i nostri concittadini, per le Forze dell'ordine che oggi sono chiamate a un compito ancora più difficile, con maggiori rischi, anche di salute, ma vogliamo la sicurezza per il futuro del Paese. Queste sono le dichiarazioni che vogliamo sentire dal Governo, e non come nemici,

Senatore Candiani, la ringrazio per aver anticipato il mio intervento e per aver esplicitato che avrei trattato questioni afferenti all'incarico istituzionale che ricopro da novembre del 2018; quello stesso incarico istituzionale per cui, spesso e volentieri - molto più spesso di quanto non si possa credere - mi debbo rapportare - come è giusto che sia - con prefetti, questori, autorità che sul territorio, rappresentando il Governo, debbono - lo garantire i diritti costituzionali ai cittadini. Ebbene, le posso garantire che, avendo sentito immediatamente chi rappresenta lo Stato, il Governo a Napoli, ho avuto la certezza di come quelle stesse persone, dal primo all'ultimo della catena di comando e non soltanto, fossero del tutto impegnate con tutte le loro energie per garantire che a Napoli, così come a Roma, a Milano piuttosto che a Torino, l'ordine democratico, che la Repubblica ha istituito dal 1° gennaio 1948, non venisse violato. Voglio anche approfittare di una singolare coincidenza, Ministro, e lo dico a voce bassa perché questo è il momento in cui bisogna ragionare, bisogna abbassare i toni, come ha fatto per esempio - l'ex sottosegretario Candiani; come ha fatto anche il rappresentante di Forza Italia Dal Mas; come, però, non hanno fatto tutti in precedenza, anche appartenenti a Gruppi che, richiamandosi alle possibilità dell'opposizione, volevano far capire quanto fossero disposti a dialogare. La senatrice Garavini ricordava come in funzione della cosiddetta legge Mancino si potrebbe sciogliere Forza Nuova. Io ricordo a me stesso che oggi è il 28 ottobre e il 28 ottobre del 1922, secondo gli storici, iniziò una marcia che poi si concluse molto tristemente per il nostro Paese, alimentando vent'anni di cancellazione delle libertà personali e sociali; alimentando un'ideologia cui tanti, che sono scesi proditoriamente in piazza a Napoli e non soltanto, si richiamano. Ora, vorrei far comprendere a tutti che è nell'interesse di chi è veramente democratico, e non soltanto a parole, richiamarsi a Gorgia, come ha fatto il senatore Dal Mas, quando ha ricordato che la politica può e deve essere in qualche modo esempio. l'esempio con cui noi dobbiamo tutti i giorni confrontarci non è tanto, o meglio non è soltanto - senatore Casini - l'esempio di chi predica in un modo, chiedendo collaborazione, offrendola e poi abbandonando l'Aula. L'esempio è quello di chi, anche occupando seggi parlamentari, ha sostenuto che l'epidemia si potesse fronteggiare con Lambrusco e salame all'aglio, perché anche questo alcuni noti parlamentari delle cosiddette opposizioni hanno avuto modo di far sapere *urbi et orbi*, approfittando - lasciatemelo dire

perché il Ministro ci ha ricordato che in questi contesti - per come anche le immagini, che sono state quasi vivisezionate, hanno potuto accertare - non soltanto ci sono stati militanti dell'estrema destra animatori di centri sociali, ma ci sono stati anche negazionisti che forse hanno tratto forza dal fatto che c'era qualcuno che la mascherina se la strappava, come se fosse la prima castrazione delle libertà individuali, perché si voleva istituire una dittatura sanitaria. Adesso quelle stesse persone hanno difficoltà a lavorare con la mascherina, anche se è l'ultimo dei fastidi. Ricordo a me stesso una parlamentare che alla Camera dei deputati, essendo affetta da gravi patologie, ha ricordato che, se la poteva usare lei, la potevamo usare tutti, a tutela, oltre che della propria dignità, anche e soprattutto del bene sacrosanto della salute che appartiene a tutti e soprattutto ai soggetti - senatore Calderoli, come lei - con difficoltà relative al fatto di essere, dal punto di vista delle difese immunitarie, più provato di altri. Lei, infatti, pochi giorni fa ha scritto qualcosa sui suoi profili *social* che a me sarebbe piaciuto far leggere a tanti suoi colleghi, perché quegli inviti provengono da altri suoi colleghi che dimostrano un grandissimo senso di responsabilità, salvo poi essere puntualmente sconfessati da chi ha

per esempio - devo dire che l'invito che ci è stato fatto - quello sì, Ministro - di potenziare la polizia postale, mi sembra doverosamente da valutare e assecondare. È stramaledettamente vero che sui *social* si realizzano inviti che in tempo reale portano decine e forse centinaia di manifestanti, che non aspettavano altro, a scendere dai Quartieri spagnoli, dalla Pignasecca di Napoli, lì dove poi ci sono stati problemi. Vorrei ricordare a tutti che a Napoli in particolar modo - e le immagini sono state chiarissime - due mezzi delle Forze dell'ordine hanno subito dei tentativi di isolamento e poi per fortuna sono riusciti a ritornare dalla parte giusta senza che si realizzasse la tragedia. Lo dico perché forse qualcuno si è dimenticato che a Genova diciannove anni fa, per una situazione che doveva essere impedita, c'è stato qualcosa di allucinante che poi rimane come un macigno sulla coscienza collettiva del Paese. Allora, proprio perché bisogna abbassare i toni e bisogna ragionare, signor Ministro, la ringrazio perché mi era sfuggito un dato era sfuggito un dato su cui vorrei che tutti quanti ci soffermassimo. A Milano, per i disordini che si sono verificati la notte del 26 ottobre, su 28 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria ben 13 risulterebbero esser minorenni. Io ho sentito dire dal senatore Candiani che, quando le manifestazioni si sviluppano soprattutto nei centri storici, si deve essere ancor più allertati per la prevenzione. Mi domando allora se per caso centri di residenza di cittadini che non sono tutelati dalla Costituzione italiana; se per caso dobbiamo ancora distinguere con un'ottica quasi classista chi è cittadino del centro storico e chi è cittadino del quartiere degradato. Forse è motivo di scandalo, e dunque di riflessione per chi vuole una politica alta, evitare che vi siano zone delle nostre città e dei nostri paesi in cui il degrado sociale sia massimo.

*(Applausi)*. È qua che io lancio una proposta, sia alla maggioranza di Governo di cui io stesso faccio parte, sia alle opposizioni tutte. Coesione significa, piuttosto che annullare le distanze e le differenze, quantomeno ridurle, far capire a chi è indietro che c'è qualcuno che sta davanti che lo sta aspettando. Ebbene, io appartengo a una forza politica che da quando è nata ed ha mandato in Parlamento suoi eletti ha chiesto a tutti loro di essere capaci di rinunciare a qualcosa delle loro indennità, perché con questo qualcosa si mandava un segnale forte a chi era meno fortunato. se noi vogliamo far capire anche in termini di ristori a chi ha partita IVA, a chi è lavoratore autonomo, a chi in qualche modo sperimenta nel quotidiano cosa sia la difficoltà del resistere, un segnale forte da parte non soltanto dei parlamentari...

mi debbo pentire per il fatto di non essere stato capace di farglielo capire, ma cerco di farglielo capire dicendolo, per cui sto concludendo. Stavo dicendo che ci sono tanti burocrati, tanti dirigenti, funzionari di pubbliche amministrazioni, tanti lavoratori dipendenti che in questi mesi non sono stati minimamente toccati dal punto di vista stipendiale. Pertanto lancio l'idea di un contributo di solidarietà, che potrebbe essere un segnale forte per quell'Italia che ha difficoltà e deve capire che si è tutti sulla stessa barca, a cominciare da chi presiede attualmente l'Assemblea.

Signor Presidente, l'intervento è un po' tardivo rispetto alle notizie di stampa già di ieri e, quindi, è notorio il fatto che abbia deciso di lasciare il MoVimento 5 Stelle.

parlamentare. Nella spiegazione più specifica ho scelto di parlarne in un'altra sede, ma quello che voglio evidenziare è che pare che tutto sia nato dalla presenza a Verona al Congresso della famiglia più volte riportato nella stampa anche nei mesi passati, ma mai si è fatto riferimento al fatto che il giorno prima fossi stata all'Aquila Film Festival, invitata a una tavola rotonda, con vari esponenti di diversi schieramenti sui temi di singolo e famiglia, tra l'altro l'altro organizzato da famiglie arcobaleno e LGBT. E questo perché erano stati già invitati più volte esponenti del MoVimento 5 Stelle e nessuno di loro ha dato disponibilità. Il particolare importante che voglio sottolineare riguarda - attenzione a questa data - il 27 maggio 2020. Da parte di un collaboratore del vice ministro Castelli per le vie brevi ricevo il seguente commento:

Non so se ci rendiamo conto della portata di questo fatto. Ma soprattutto, a parte gli ostacoli che ho incontrato sia sul territorio da parte di alcuni colleghi che qui nelle Aule

di non aver agito in maniera congiunta per le esigenze che riguardano la Sicilia. Spesso mi si è detto che sarei passata alla Lega, non farò, e ho già spiegato ai colleghi per quale motivo. Ma devo ammettere che vedo più attenzione alla Sicilia da realtà che dovrebbero apparentemente essere lontane rispetto a a quelle che dovrebbero essere vicine. Siamo stati 53 parlamentari eletti in Sicilia. Quali i temi lasciati in sospeso? Solo l'emergenza sisma;

il mancato rientro dei docenti esiliati. Inaccettabile è la chiusura del Ministro dell'istruzione all'istanza di rientro di docenti da anni lontani dai propri cari, dovendo sostenere spese di vitto, alloggio, trasporto e altro ancora, di cui il Ministro non si fa carico. Non è un problema nato oggi, ma il Governo e il MoVimento 5 Stelle, nonostante quest'ultimo avesse promesso in campagna elettorale un concreto intervento, non hanno mostrato alcuna sensibilità sul tema. Occorre riordinare tutto il processo di mobilità, stabilizzazione e assunzioni. Come ebbe a dire

dello spettacolo viaggiante. C'erano varie sigle sindacali, le ho incontrate e ho parlato con molti e sono entrato nelle specifiche questioni. Ho conosciuto molte persone dignitose che mi hanno raccontato il loro problema. Da marzo